per chiedere alla Presidenza del Senato di sollecitare la ministra della giustizia Cartabia a venire con urgenza in quest'Aula per una comunicazione del Governo sulle torture inflitte ai detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere da personale della polizia penitenziaria. Presidente, ho usato a ragion veduta il termine tortura, perché solo così riesco a definire, ai sensi della legislazione italiana e delle convenzioni internazionali, i fatti di cui siamo venuti a conoscenza, non da voci o indiscrezioni, ma attraverso le immagini incontestabili registrate dal circuito di sicurezza del carcere. Abbiamo appreso che tali violenze si ripetevano da tempo

per la necessità del Senato di capire, dobbiamo sentire il Governo per cercare vie urgenti di intervento, parlamentare e anche legislativo. È questo il senso della richiesta alla ministra Cartabia di venire al più presto in Aula per comunicazioni del Governo. Negli ultimi decenni, signor Presidente, il Parlamento ha perso molta della centralità che la Costituzione gli ha assegnato nell'ordinamento, ma su fatti come quelli emersi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non sarebbe concepibile che il Parlamento non si esprimesse con tutta la forza che la Costituzione gli attribuisce. È per questo che è urgente che le comunicazioni del Governo vengano portate in quest'Aula nel più breve tempo possibile. *(Applausi)*.

Tenuto conto che avevamo previsto il voto per il disegno di legge costituzionale, che prevede una maggioranza qualificata, intorno alle ore 11, se i colleghi sono d'accordo, non volendo limitare

tenuto conto che, per via dei tempi della sanificazione, ieri sera non si sono potuti svolgere gli interventi di fine seduta,

che l'ha determinata, poiché era da sempre un nostro importante punto di vista quello di consentire

parziale e lo abbiamo anche espresso in occasione della precedente lettura in Senato, perché avremmo preferito una riforma che modificasse anche l'elettorato passivo, equiparandolo

della nuova composizione complessiva del Parlamento sarà del Senato, quindi si ridurrà ancora di più la presenza di giovani nelle nostre Camere. Questo avrebbe dovuto spingerci a pensare ad una riforma più complessiva dell'elettorato, sia attivo che passivo, del Senato.

la funzione del Senato italiano, perché non vota il bilancio e non vota la fiducia al Governo. Pensiamo, quindi, che vada approvato e salvaguardato l'impianto perché comunque consente di parificare l'elettorato attivo a quello della Camera, quindi è un passo in avanti e come tutti i passi in avanti deve essere sostenuto, ma crediamo anche che sia una riforma incompleta.

qualcuno si è stancato di sentirci dire sempre le stesse cose, ma nel 2016 Matteo Renzi, allora Presidente del Consiglio, propose una riforma che poteva avere tante criticità e fu bocciata dagli elettori - quindi rimane quello

del no era stato chiamato ad offrire una proposta alternativa; qualcuno diceva che con pochi articoli si potevano fare quegli interventi che erano previsti nella riforma bocciata il 4 dicembre 2016; quei pochi articoli non li abbiamo più visti e i problemi che cinque anni fa

saranno ancora più pesanti nella prossima legislatura, nella quale un minor numero di parlamentari si dovrà confrontare con una situazione istituzionale immodificata, quindi sempre con due Camere che legiferano, sempre con il meccanismo della fiducia

parlare oggi di riforme spezzatino - che noi siamo i primi a condannare - non ha tanto senso, perché ricordiamo bene quale fu il giudizio della maggior parte delle forze politiche nel 2016, quando quel *referendum* poteva cambiare le cose.

cui l'uscita dalla pandemia catalizzerà l'attenzione della vita parlamentare e dei lavori parlamentari, come vediamo anche ora con i tanti provvedimenti legislativi che sono all'attenzione delle Commissioni e che quindi arriveranno in Aula nel periodo estivo.

nell'ultimo anno. Mi riferisco soprattutto, ad esempio, al tema del Titolo V e al rapporto tra Stato e Regioni, che sarà un altro di quei temi che il Parlamento non si potrà sottrarre dal rivisitare. È del tutto evidente, infatti, che quello è veramente il nocciolo duro delle questioni istituzionali del nostro Paese. Abbiamo assistito ad una difficoltà di dialogo negli ultimi mesi tra Stato e Regioni, soprattutto nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, che ancora oggi grida vendetta. C'è bisogno, quindi, soprattutto sul tema della legislazione concorrente, di mettere nel tempo la parola "fine" per lasciare allo Stato e alle Regioni ambiti di azione chiari ed evidenti, evitando contrapposizioni che poi diventano elementi di contrapposizione che creano sfiducia nei cittadini che non sanno più qual è il soggetto istituzionale di riferimento. Apprezziamo l'impianto di questa riforma e la voteremo con convinzione, ma c'è in noi un rammarico, perché sarebbe stato più giusto un provvedimento che rivedesse non soltanto le soglie le soglie di età dell'elettorato attivo, ma anche e soprattutto le soglie di età dell'elettorato passivo. Auspicando che si possa poi mettere mano al sistema istituzionale in maniera più complessiva e più adeguata alle esigenze di uno Stato moderno e dei cittadini,

Signor Presidente, vorrei cominciare questa mia breve dichiarazione di voto con una riflessione che Aldo Moro fece a proposito degli avvenimenti del 1968. La cifra di quel tempo imprendibile eppure così denso, era data dall'affacciarsi sulla scena pubblica di un nuovo soggetto sociale fino ad allora prigioniero di una condizione sotto tutela: i giovani. Moro parlava dell'urgenza di un tempo nuovo; è una nuova umanità che vuole farsi. Oggi il voto generalizzato a diciotto anni deve essere inteso come l'inizio di un tempo nuovo, ma c'è bisogno di una consapevolezza piena di questa scelta. Non è un adattamento costituzionale dovuto a un'esigenza di simmetria elettorale; è una scelta politica di responsabilizzazione di un soggetto sociale, appunto i giovani, i giovani, senza più distinzioni tra loro, padroni delle proprie scelte e del proprio futuro. Il voto di oggi segna un passaggio cui la politica, noi, dobbiamo essere all'altezza di questa scelta. Dobbiamo essere credibili agli occhi di chi si affaccia per la prima volta al voto e, quindi, alla partecipazione più alta di una comunità democratica. La credibilità è figlia della serietà e della responsabilità. Se siamo consapevoli del senso del voto che stiamo per dare, questo ci impegna a essere politicamente seri allora, possiamo dire che questo voto di modifica costituzionale è un impegno che noi tutti in questo Parlamento ci assumiamo e che consegniamo a chi ci dovrà e ci saprà giudicare. Il voto del Gruppo per le Autonomie sarà favorevole.

Fratelli d'Italia dal percorso iniziato alla Camera è convinta che questa sia una riforma giusta a metà. Da sempre parliamo di questa legge. La destra lo fa non da oggi, ma da quando Giorgia Meloni, allora Ministro della gioventù, fu la prima a portare all'attenzione dell'Aula la necessità del coinvolgimento dei giovani nella vita politica, con l'abbassamento - in quella proposta di legge si Fratelli d'Italia, però, non si è mai sottratta alle sfide delle riforme costituzionali, seppure in questa versione puntuale mantenendo - noi sì - quella visione organica che è propria culturalmente della destra. Sul tema delle riforme costituzionali, ad esempio, in questa legislatura siamo stati determinanti e siamo sempre stati componente necessaria all'approvazione della riforma che ha portato alla riduzione dei parlamentari, ed è bene ricordare che anche dall'opposizione abbiamo votato per il taglio dei parlamentari che senza il nostro voto non si sarebbe realizzato. Allo stesso modo, vogliamo essere decisivi e determinanti anche su questa riforma, così come sulle tante altre sfide di modernizzazione del nostro impianto ordinamentale. Ciò non ci impedisce di rilevare con rammarico che avremmo voluto che vi fosse quell'equiparazione che abbiamo provato a inserire tanto alla Camera quanto al Senato con emendamenti puntuali per affermare che il principio che, se puoi votare, alla stessa età puoi anche essere votato; se hai la capacità di scegliere chi ti rappresenta, puoi essere anche tu quello che rappresenta gli interessi diffusi e il futuro della nazione, dando così voce e protagonismo ai giovani. Su questo credo che non accettiamo lezioni da nessuno perché la destra è sempre stata nella storia avanguardia in questo senso. Certo, siamo consapevoli che quella dei giovani è una categoria che sembra inspiegabilmente esclusa dalla vita politica parlamentare, tanto alla Camera, quanto al Senato. È una categoria esclusa soltanto in Italia perché, invece, nel resto dell'Europa i diciottenni partecipano direttamente alla rappresentatività parlamentare. È così in Danimarca, Finlandia, Germania, Olanda e in altri Paesi europei. Se vogliamo però che i giovani rappresentino in questo Parlamento anche quel pezzo di società nazionale e quindi il futuro, la speranza e l'ambizione della nostra Nazione, non basta questa piccola riforma, se non possono essere loro stessi a rappresentare quello spaccato di società. Non pensate che in questo momento, se in Aula ci fossero ragazzi di diciotto o diciannove anni, sarebbero stati in grado di rappresentare il disagio, le ambizioni e le preoccupazioni dei propri coetanei? Elementi di cui spesso, proprio in questa Aula, anche in provvedimenti recenti non si è tenuto conto. Alla luce soprattutto di un'epidemia, così devastante ed impattante proprio sui giovani, è evidente che oggi i media e i *social media* accelerano i processi di comunicazione, di informazione di formazione delle coscienze e quindi anche il coinvolgimento dei più giovani nella vita politica si concretizza meglio rispetto a quelli che probabilmente erano gli intendimenti ai tempi della scrittura della Costituzione. Rimane però un *vulnus* rispetto alla possibilità, come abbiamo detto, di scegliere rispetto al proprio destino. Sono tanti i temi e i provvedimenti varati i cui effetti si sono scaricati proprio sui giovani. Pensiamo, ad esempio, alla riforma delle pensioni avvenuta qualche tempo fa. Scelte ricadute sulle future generazioni senza che queste generazioni abbiano potuto dire la propria su quelle scelte che si trovano a pagare. Oppure, per fare un riferimento recente, ricordo gli importanti scostamenti di bilancio che abbiamo votato in Assemblea per rispondere alle esigenze della pandemia. Sono ipoteche sul futuro delle giovani generazioni di cui non si è tenuto conto e che forse avrebbero potuto dire la propria qualora tali risorse fossero state utilizzate per le infrastrutture e per lo sviluppo economico, anziché sprecate per *navigator*, *cashback* o per il reddito di cittadinanza. questo appello anche nell'*iter* parlamentare, ma va registrato che, proprio qui in Senato, la politica della maggioranza di allora si è arenata e si è tirata indietro su quello che il Senato aveva fatto, con l'equiparazione anche dell'elettorato passivo. Fratelli d'Italia voterà a favore della riforma al nostro esame perché non ci siamo mai tirati indietro nelle sfide di rinnovamento a cui abbiamo sempre approcciato con una visione organica. che non si può prescindere da un presupposto fondamentale che va introdotto nella Costituzione accanto alla riduzione del numero dei parlamentari e alla maggior partecipazione dei giovani: l'elezione diretta del capo dello Stato. Ciò per rimuovere tutte quelle barriere che il nostro ordinamento ha alla piena partecipazione dei cittadini alla vita politica, che per noi significa rispetto del voto dei cittadini, che non è un assegno in bianco con cui i partiti possono fare quello che vogliono o quello che gli conviene in quel dato momento storico. Tutto ciò nella logica della difesa delle Istituzioni e di un impegno al rinnovamento delle stesse, guidati, come siamo sempre, solo da un unico interesse, quello nazionale e quello degli italiani.

Vedo il Ministro dei rapporti con il Parlamento, che ha anche la delega alle riforme, e mai, come in questo giorno, la sua presenza è davvero coerente con il percorso che è stato fatto. Dovremmo infatti anche ricordare

e di continuo approfondimento tra i membri delle due Commissioni di Camera e Senato per provare ad arrivare a dare una risposta che raccogliesse le esigenze che i parlamentari stavano portando sul campo rispetto a questo aspetto

diciamo una cosa molto chiara: pareggiamo, dicendo a tutti quei ragazzi compresi in ben sette fasce di età, dai diciotto ai venticinque anni, che la politica ha bisogno di loro e ha bisogno della loro capacità di scegliere. Questo dà a noi una responsabilità. Ieri ho sentito in discussione generale che qualcuno sottolineava il fatto che ci sia un impoverimento della conoscenza, del senso civico italiano, delle nostre regole, delle nostre leggi, del funzionamento delle istituzioni. Ebbene, non possiamo lanciare noi l'allarme da questi banchi; noi dobbiamo trovare la soluzione e la risposta

proprio dei più giovani, sui temi che a loro stanno a cuore: i temi dell'ambiente e dei diritti. I ragazzi ci sono nelle piazze e vogliono partecipare. E allora aiutiamoli noi,

Questo può aiutare ad aumentare anche la partecipazione al voto, perché spesso, dopo le elezioni, ci trasformiamo anche noi in commentatori e raccontiamo come poi il partito più forte sia spesso, troppo spesso, quello dell'astensionismo. Allora il fatto di voler coinvolgere questa fascia d'età anche per quanto riguarda il voto al Senato, garantendo loro questo tipo di diritto, può essere un ulteriore tentativo di dare una risposta a tale

giornata, perché è come se il legislatore oggi rispondesse a loro, rispondesse a queste istanze. Aggiungo un elemento, che indubbiamente è politico, perché la riflessione che è stata fatta nelle Commissioni di Camera e Senato dal relatore Parrini, che ringrazio per il lavoro che ha svolto, di grande attenzione, insieme a tutti i membri della 1a Commissione della 1a Commissione del Senato, è stata una riflessione profonda su questi bacini elettorali, differenti fino a oggi, che hanno spesso portato a una differenza di composizione numerica delle maggioranze tra Camera e Senato, che spesso ha messo in difficoltà la nostra attività nel portare avanti le istanze e nel dare stabilità al Paese. Non è detto che in questo modo si risolva tutto, ma indubbiamente il fatto di garantire due bacini elettorali identici, almeno dal punto di vista anagrafico, che quindi andranno a scegliere i membri di Camera e Senato esattamente nello stesso modo, con due schede differenti, ma votati da tutti, tutti, forse potrebbe aiutare a migliorare lo stesso funzionamento delle nostre istituzioni. Anche questo andrebbe spiegato, perché abbiamo la necessità che le nostre istituzioni e la modalità con cui lavoriamo vengano conosciute. Spesso noi risultiamo semplicemente quelli nel palazzo, con pochi contatti all'esterno. In realtà magari qui dentro si cerca spesso di fare un lavoro che possa portare avanti le istanze che arrivano da fuori. Io penso che questa sia un'opportunità ulteriore che noi oggi, come classe politica, dobbiamo cogliere;

La politica ha una serie di temi su cui interrogarsi: sulla sua capacità di comunicare quello che fa, sulla capacità di dimostrare il lavoro che si fa in queste Aule, sulla capacità di raccontare la difficoltà del processo legislativo nello scambio, anche nello scontro, nella voglia di trovare la sintesi. Anche queste sono opportunità che abbiamo, dicendo ai ragazzi più giovani che offriamo - perché ci crediamo - una carta in più che dà loro un elemento - uso questo termine - di cittadinanza. È come se dicessimo che vogliamo garantire un'ulteriore protagonismo della vita civile proprio per tutti i più giovani. Presidente, parlo con grande serenità perché ho sentito chi ha parlato di riforma spezzatino; lo ricordava anche prima il senatore Grimani: ricordava processi di riforma che sono stati fatti in maniera più complessa e che poi magari non hanno portato a casa i risultati che molti, invece, speravano di poter ottenere. Vediamolo, sì, come un piccolo passo, ma vediamolo come un passo che compie il Parlamento

che alle prossime elezioni potranno votare per tutti e due i rami del Parlamento. la riforma che approviamo oggi in modo definitivo è certamente un segnale importante importante nei confronti dei giovani, come lo è stato il riferimento nell'altra riforma - per me, devo dirlo con franchezza, molto più importante - che abbiamo approvato in prima lettura

che chiedevano ai decisori politici di assumersi la responsabilità della loro vita, quindi di scelte concrete per contrastare i cambiamenti climatici, di scelte concrete per il loro futuro,

Perché dico che è nella responsabilità della politica? Perché spetta a chi poi deve dare un volto diverso della politica, dell'assunzione di responsabilità e dell'interesse generale; a chi deve lavorare per modificare lo stato delle cose e dare ai giovani delle prospettive vere. Il problema dei giovani oggi è anche quello del futuro

al Senato il problema delle differenze degli esiti elettorali, che ha accompagnato un po' tutta la storia del nostro Paese,

giustamente diamo la possibilità di poter esercitare il loro elettorato attivo anche per il Senato, in molte Regioni potrebbero non veder rappresentato il voto che esprimono per la prima volta. Questo è un problema che sta tutto davanti a noi.

non abbiamo più affrontato il tema della modifica della legge elettorale per avere un sistema che possa far sì che non ci sia una compressione, con la riduzione del numero dei parlamentari, della rappresentanza politica e territoriale. È una questione che, a maggior ragione nel momento in cui interveniamo per allargare l'elettorato attivo al Senato, si pone con forza, perché non è detto che possano

l'allargamento dell'elettorato attivo ai diciottenni per il Senato non risolve il problema

Noi, al contrario di Italia Viva, siamo stati assolutamente d'accordo ad eliminare da questa riforma la modifica dell'elettorato passivo. Lo dico perché non pensiamo e non vogliamo pensare che questa riforma dovesse essere soltanto l'anticamera di fatto dell'eliminazione del Senato o di

rimangono però davanti a noi non risolte le questioni che ho posto e che noi continuiamo a rimuovere. La riduzione dei parlamentari, tuttavia, pone con forza una questione di equilibrio del sistema, oltre alla questione del pluralismo del pluralismo politico e della rappresentanza territoriale. Spero in ogni caso che, anche dopo l'approvazione finale di questa riforma, finalmente a tutto questo, affrontando una volta per tutte in modo serio la questione della legge elettorale per tentare di ridare rappresentanza

Certamente dunque questa riforma è positiva, perché propone e permette un allargamento della partecipazione, ma rimane davanti a noi la questione molto seria del del pluralismo politico e della rappresentanza.

spiegando perché noi non ci siamo associati al coro pressoché unanime a favore della riforma che stiamo approvando. Voglio aggiungere però qualcosa. Ci troviamo di fronte a uno dei provvedimenti che ci erano stati promessi quando, l'anno scorso, si è votato per la drastica riduzione del numero dei parlamentari.

Nel 1963 si stabilì il numero fisso di 315 senatori eletti, cioè uno ogni 98.000 elettori. Nel 2018, delle ultime elezioni, il numero di elettori per ogni senatore è passato da 98.000 a 148.000 per via dell'aumento della popolazione italiana. Di fronte a questo, si è pensato di ridurre il numero dei senatori, portandolo a 233.000 elettori per ogni eletto, per cui siamo passati da 98.000 nel 1963 a 233.000 con le precedenti riforme.

di giovani, che avranno molto meno potere di quello che avrebbero avuto prima della riduzione del numero dei parlamentari, quando avrebbero potuto votare per un adeguato numero di deputati. *(Applausi)*. Se questa è la compensazione, siamo completamente fuori strada.

ha cambiato Gruppo due volte, per il nobile fine di aiutare a dar vita al Gruppo degli europeisti, che era fatto tutto da cambiatori di casacca, allo scopo di sostenere il terzo Governo Conte. *(Applausi)*. Se l'esempio viene da lì, l'esempio viene da lì, dove andiamo a finire? Peraltro, lo stesso Enrico Letta divenne Ministro (una delle tre volte che lo è stato) prima di essere mai eletto a qualsivoglia carica: è stato particolarmente dotato, perché ha fatto tre volte il Ministro senza neanche essere mai stato eletto consigliere comunale, ben lontano dall'essere deputato. Il primo Governo in cui fu Ministro fu il primo governo D'Alema, che nacque grazie al cambio di casacca di molti deputati e senatori da Rifondazione Comunista, da Forza Italia e persino da Alleanza Nazionale. *(Applausi)*. Allora riuscirono a mettere insieme degli eletti di Rifondazione Comunista e di alleanza Nazionale pur di fare un Governo, pur di fare Enrico Letta ministro, che era un traguardo atteso dalla fine della guerra. Non basta: Enrico Letta è stato anche Presidente del Consiglio (lo ricordiamo bene), anche con il nostro voto, ahinoi. Quel Governo nacque da una maggioranza originata dal premio di maggioranza ottenuto dal Partito Democratico

ma non vanno a votare, magari perché vedono poca serietà e, conoscendo i *social media* meglio di qualunque altra categoria d'età, vorrebbero che la politica avesse un livello diverso e non fosse quella dei *like.* Ricevere dei *like* è una cosa, governare un Paese è un'altra e i giovani lo sanno bene. *(Applausi)*. Se si fanno le riforme costituzionali dei *like,* i primi a capire che è una fregatura sono i giovani. questo modo creiamo una premessa. Equiparando l'età per votare al Senato e alla Camera, rendiamo meno giustificabile il bicameralismo. Ora, il bicameralismo a qualcuno piace e a qualcuno non piace, ma ricordo che il 4 dicembre 2016 gli italiani hanno respinto il sostanziale monocameralismo introdotto dalla riforma Renzi-Boschi e

del giorno dopo, dicono: chi se ne importa. Il comportamento serio sarebbe un altro, ma, per raccattare qualche consenso, facciamo anche così. Dovrebbero sapere che la Costituzione

stabilità democratica e alle potenze straniere che cercano di infilarsi nel nostro territorio (parlo del regime del Partito Comunista cinese), comprando aziende, persone e *media*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi tutti sappiamo che i Padri costituenti, allorquando decisero di dare alla democrazia italiana la struttura bicamerale che ben conosciamo, erano anche ben consci che la democrazia rappresentativa postula un problema, che non definirei di difficile, ma quasi di impossibile soluzione. è quello di garantire, tramite il sistema elettorale, che i rappresentanti eletti siano la fedele proiezione dell'elettorato, di modo che in queste Aule siedano,

il metodo elettorale per l'una e l'altra Camera, in modo da ottenere due diverse fotografie del Paese, che, una volta sovrapposte, dessero una rappresentazione maggiormente ricca di dettagli. La *ratio*, dunque, della differenza tra l'elettorato attivo alla Camera e al Senato non risiede, come chiarirò

tra i due elettorati era di soli quattro anni. Tutti sappiamo che la maturazione della persona subisce un'accelerazione man mano che si cresce: tanta è la differenza in termini di maturità tra un dodicenne e un sedicenne, ma assai poca, direi nulla, è tra un ventunenne e un venticinquenne. Quindi, la *ratio* iniziale era ben diversa

Camere idonea a controllare l'altra. Costantino Mortati, tante volte citato (chissà quante volte letto), ci ricorda che vi è differenza...

Costantino Mortati ci ha spiegato che vi è differenza tra Costituzione formale e materiale e la Costituzione materiale che oggi integra la Costituzione formale è diversa. Ormai siamo di fronte a un bicameralismo alternato; specialmente con i decreti-legge, vediamo che i provvedimenti partono una volta dalla Camera, un'altra dal Senato. Solo per i disegni di legge di iniziativa parlamentare ritroviamo quel bicameralismo.

E se valutiamo anche la modifica di fatto del nostro assetto costituzionale, ci rendiamo conto ulteriormente che non vi è più la necessità di tenere distinta l'età degli elettori della Camera e del Senato. Per quello che ho detto, allora, non è esatto forse intendere questo provvedimento come un'apertura ai giovani, perché bisogna far loro spazio. Il problema non è questo,

non può essere considerato isolatamente, come fine a se stesso. Esso si deve accompagnare a un'operazione ben più ampia

Qual è la via per migliorare la coscienza politica, sociale e civica degli italiani? I *social network* - non lo nascondiamo - non ci stanno aiutando. Uno dei passaggi fondamentali per questa presa di coscienza risiede nell'esempio che noi per primi dobbiamo dare. L'epoca delle contrapposizioni ideologiche, in cui eravamo nemici, risale ad almeno settant'anni fa. fa. Oggi siamo espressione di una democrazia che tenta disperatamente di diventare matura, in cui non ci sono nemici, ma avversari, che si confrontano sulle idee. Una vera democrazia, affinché ognuno di noi sia davvero rappresentante del popolo, chiede e impone una mediazione.

sono portatori di altre idee che non possiamo ignorare e sappiamo - e l'abbiamo dimostrato con i fatti - che, se siamo veramente democratici, per portare un provvedimento all'approvazione è necessaria la mediazione. Se diminuiamo l'età dell'elettorato a diciotto anni, ma continuiamo a spaccarci

Dobbiamo essere all'altezza del provvedimento che stiamo approvando. Dobbiamo mostrare agli italiani come ci si comporta, quando si è consci

perché, se continuiamo a procedere così, continueremo a rivolgerci a un elettorato che, magari novantenne, rimarrà immaturo, perché non adeguatamente informato

ripercorrerò quanto sostenuto dai colleghi che non voteranno favorevolmente a questa riforma apparentemente minimale dalla Costituzione, ma niente affatto irrilevante, riportando all'attenzione di quest'autorevole Assemblea alcuni passaggi dei lavori preparatori della 1a Commissione di questo ramo del Parlamento. Si è detto che i Padri costituenti avevano previsto una differente età di elettorato per le due Camere e che questo qualcosa vorrà pur dire. Nell'affrontare il tema della diminuzione della soglia per accedere all'elettorato attivo a diciott'anni anche per il Senato, non si può non considerare il mutato contesto socio-culturale del Paese rispetto alla stagione costituente del 1946-1947, i cui lavori devono costituire un imprescindibile punto iniziale. Le ferite della guerra e della fase istituzionale che precedettero il dibattito sulla Costituzione consigliarono i costituenti di prevedere elementi differenziali nella composizione su base anagrafica del corpo elettorale,

attivo di Camera e Senato, com'è noto, era pari a quattro anni, quando la Costituzione entrò in vigore. Tuttavia, nella legge n. 39 del 1975, che fissava il compimento della maggiore età a diciott'anni rispetto ai ventuno precedentemente previsti, tale differenza è stata raddoppiata e dunque si sono amplificati gli effetti delle scelte dei costituenti, in un periodo peraltro di maggiore progresso e scolarizzazione. La circostanza che la legge ordinaria, che perseguiva tutt'altre finalità, abbia conseguito un simile effetto distorsivo e di scoordinamento tra i commi 1 degli articoli 48 e 58, va necessariamente sanata, perché priva di giustificazione e senza uguali nelle democrazie contemporanee. Si è detto: non voteremo una riforma fatta - cito testualmente - «a spizzichi e bocconi». Allora, ditelo che volete abolire una delle due Camere. Era il 1985 quando la Commissione Bozzi, nella sua relazione conclusiva, auspicava per la prima volta la fissazione dell'elettorato attivo al Senato al conseguimento della maggiore come per tutti gli altri diritti civili e politici. Diverse ipotesi di riforme istituzionali hanno annoverato l'abbassamento dell'elettorato attivo, sino al fallimento della riforma Renzi-Boschi. L'esito del *referendum* del 4 dicembre 2016 e con esso l'abbandono - voglio sperare - di ogni ipotesi di elezione indiretta del Senato e, più in generale, delle variegate proposte volte a introdurre una differenziazione strutturale o funzionale tra le due Camere hanno dato luogo a una limitazione del principio di uguaglianza del cosiddetto voto in entrata che, sebbene fissato da norma di rango costituzionale e, quindi, non di per sé illegittimo, non risulta essere meno indigesto alla luce dei princìpi democratici. Concedendo la facoltà di voto a determinate categorie anagrafiche di cittadini ritenuti presuntivamente più capaci e idonei, si lede la libertà di scelta del corpo elettorale e, quindi, la stessa libertà di voto. I *referendum* del 2006 e 2016 hanno insegnato a chi ha voluto coglierne la lezione che ulteriori tentativi di procedere a riforme costituzionali complessive sono destinati al fallimento per la difficoltà di far comprendere, soprattutto durante la campagna referendaria, le linee di fondo di un progetto ampio. Così, il legislatore, quindi noi, è stato spinto verso l'adozione del metodo opposto, ovvero riforme puntuali, dando per altro seguito alla *ratio* con cui fu scritto l'articolo 138 della Costituzione, ampiamente riconosciuto dalla dottrina. Si è detto: i giovani non sanno chi sia il Presidente della Repubblica, come possiamo concedere loro il diritto di voto? La menomazione del diritto di voto è in danno proprio ai cittadini titolari di interessi meno contingenti e che perciò tendono naturalmente a privilegiare uno sguardo rivolto al futuro, con la conseguenza di un'elevazione progressiva dell'età dell'elettorato mediano derivante dall'invecchiamento della popolazione che, com'è noto, si registra in tutta Europa e, in particolare, in Italia.

nel procedimento legislativo meccanismi e incentivi volti a incoraggiare il prevalere di una visione lungimirante e di lungo periodo rispetto all'attuale dominio della logica del contingente, come si fa in Finlandia con la Commissione del futuro, da tempo operante presso il Parlamento di quel Paese. che bello sarebbe se prevedessimo un Ministero per il futuro. Inoltre, per effetto della disciplina costituzionale vigente sull'elettorato attivo si continua a differenziare la composizione di Camera e Senato con una differenza di quasi 4 milioni, accentuando così il rischio di orientamenti politici diversi tra i due rami del Parlamento e rendendo più difficile il funzionamento sia del sistema bicamerale sia della forma di Governo parlamentare. un rischio che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2017 di illegittimità sul cosiddetto Italicum, ha posto in evidenza, suggerendo al contempo una soluzione:

possiamo estendere il monito non esclusivamente al sistema elettorale, ma all'assetto bicamerale, se non all'intero sistema costituzionale. Quindi, l'omogeneizzazione delle basi elettorali di Camera e Senato gioverebbe alla funzione di Governo. Governo. Si può affermare, allora, che la riforma in esame avrebbe il pregio non banale di coniugare in una certa misura i valori di rappresentanza e governabilità, spesso in contrasto tra di loro. Si è detto: ci asterremo perché non vogliamo che i giornali ci dicano che siamo contrari ai giovani. Colleghi, quando si discorre di istituzioni democratiche, la gioventù non può essere sbandierata come un valore in senso assoluto, né tantomeno esecrata in quanto tale, ma dev'essere semplicemente considerata alla luce dei principi costituzionali. Si tratta di una riforma assolutamente opportuna, resa necessaria dalle evoluzioni sociali, culturali e istituzionali intervenute nel tempo al fine di porre rimedio agli effetti distorsivi della rappresentanza democratica che emerge dall'attuale disciplina. Intendiamoci, però: l'acclarata disaffezione alla politica delle nuove generazioni è un fenomeno che non si elimina *sic et simpliciter*, garantendo ai giovani la possibilità di votare anche al Senato; occorre oggi adottare una prospettiva di più larghe vedute, recuperando la partecipazione dei giovani alla politica, attraverso forme di rappresentanza nuove e più confacenti al mutato contesto sociale (penso, ad esempio, alla democrazia digitale). Nella fase attuale, caratterizzata da una certa crisi degli istituti classici di democrazia, la conservazione dell'articolo 58 della Costituzione rischia solo di contribuire a incrementare il divario tra popolo e votanti, indebolendo la sovranità affermata dall'articolo 1 della Carta in relazione al profilo della volontà popolare. Per queste ragioni, ribadisco il voto favorevole del gruppo del MoVimento 5 Stelle al disegno di legge costituzionale

Presidente, onorevoli colleghi, non voglio sottrarmi al dovere di manifestare le mie perplessità su questo modo di procedere per attuare importanti riforme costituzionali con una parcellizzazione, a mio avviso, molto pericolosa. Il provvedimento in esame, modificando il requisito anagrafico dell'elettorato attivo per il Senato, rischia infatti di portarci nella direzione di un preciso disegno non pienamente svelato in quest'Aula, che si potrà compiere nella prossima legislatura, con il superamento del bicameralismo perfetto. riforme, a mio avviso, è sbagliato, come lo sono questi interventi, parcellizzati e fatti con il bisturi. Attuare la lenta erosione delle differenze tra Camera e Senato potrebbe portare a compiere l'altro passo, passo, l'equiparazione dell'elettorato passivo già nella prossima legislatura, come ho detto, fino a giungere poi all'inevitabile conclusione dell'inutilità del Senato, ormai ridotto a una seconda Camera. L'Assemblea costituente, come tutti sapete, si soffermò a lungo sulla questione del bicameralismo, operando la scelta di quello perfetto, con le disposizioni necessarie a creare differenze significative tra i due rami del Parlamento. Si ritenne infatti di differenziare il sistema elettorale delle due Camere, uno su base regionale, l'altro su base nazionale, e l'elettorato attivo e passivo dei due rami del Parlamento, in base al requisito dell'età. Secondo me, tutto questo adesso va tutelato e non modificato. Esprimendo un voto favorevole sul provvedimento sarete complici di un disegno più ampio, non chiaramente esplicitato, volto a sopprimere la Camera alta, il Senato della Repubblica italiana, proprio nell'Italia che ha visto nascere il *senatus romanus*.

Tuteliamo la Costituzione, perché questa riforma rischia di essere l'anticamera del monocameralismo. In conclusione, non si intacchi il punto di forza del bicameralismo paritario, che risiede nella valorizzazione e non nella compressione delle differenze fra i due rami del Parlamento. Vi invito pertanto a valutare il provvedimento alla luce del pericoloso disegno che si sta configurando, che, a mio avviso, è insensato e contrario ai principi costituzionali, perché mina

mi associo a queste ultime parole che ho ascoltato dal collega Auddino, perché - attenzione la politica *in extremis*, in prossimità del *referendum* costituzionale, aveva garantito sul proprio onore che sarebbero stati posti in essere dei rimedi: riforme costituzionali, modifiche legislative ordinarie, modifiche dei Regolamenti parlamentari, segnatamente del Senato, prima di dare poi avvio a ulteriori riforme. Ebbene, nemmeno la legge elettorale è stata rivisitata, sebbene l'allora segretario del Partito Democratico Zingaretti avesse esultato per il raggiungimento di un accordo su un testo base. Senza quelle modifiche, stiamo regalando ai diciottenni un giocattolo rotto, perché il Senato della Repubblica non potrà funzionare; con le attuali norme, stiamo regalando loro un *bluff*, un giocattolo rotto. E allora, se sul loro onore avevano promesso quelle modifiche, ora con quale onore e con quale coraggio chiedono ancora fiducia? Coloro che disonorano la propria parola non hanno diritto ad aver fiducia, finché non ripristinano correttamente e non onorano la propria promessa. In base a quale mandato stiamo picconando le istituzioni della Repubblica, demolendo il bicameralismo paritario? In base a quale mandato ci crediamo novelli Zeus di questa ricostruzione, che è una demolizione? io voterò contro, non per un partito o per un Gruppo; io voterò contro per la mia onorabilità personale e perché non voglio essere complice di quest'ulteriore malefatta coperta. Guardate che di questa vicenda non hanno parlato neppure i necrologi della gazzetta salentina. Stiamo parlando di qualcosa che nessuno conosce e le cui conseguenze tutti patiranno. Se ci fosse stato un dibattito pubblico - e quindi un mandato - avreste avuto ragione; ma avete torto e siete un *falsus procurator*, perché non avete alcun titolo a modificare le fondamenta della Costituzione. Io voterò contro, almeno nel mio nome.

intervengo non solo per sottoscrivere la richiesta del senatore Zanda di avere qui il Ministro della giustizia, ma per mettere in evidenza il fallimento della politica. Ancora una volta abbiamo dovuto attendere che la magistratura si muovesse; eppure, da queste Aule sono partiti atti

tra domenica 5 e lunedì 6 aprile 2020. Si chiedeva al Ministro di sapere quali fossero effettivamente i fatti avvenuti in quella notte e cosa stava accadendo a Santa Maria Capua Vetere, perché già i giornali e i *social* riportavano fatti gravissimi. Ebbene, non abbiamo ricevuto alcuna risposta dalla politica: il Parlamento chiede, ma il Governo non risponde e la magistratura deve intervenire. Quindi, sottoscrivendo la richiesta del collega, anch'io faccio appello affinché, almeno adesso, in estremo ritardo, il Ministro si presenti a dare ragione di questi fatti gravissimi.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo Fratelli d'Italia si unirà alla richiesta avanzata dal senatore Zanda atta a far

Chiediamo altresì che il Ministro venga in quest'Aula a riferire non soltanto su quei fatti ma sulla situazione che, purtroppo, riguarda i nostri penitenziari.

da lei non me lo sarei aspettato, perché è un uomo molto pagato: è veramente una caduta di stile, e chiedo quindi che vengono porte le scuse nei confronti del 99 per cento degli appartenenti alla Polizia penitenziaria che svolgono il loro dovere nei nostri

carceri e sezioni date alle fiamme, agenti insultati e aggrediti, agenti di Polizia penitenziaria finiti all'ospedale. Su tutti questi fatti chiediamo al Ministro di sapere

volontà di fare una critica o dare una diversa interpretazione dei fatti. Mi associo invece a quanto ha chiesto il senatore Zanda, perché, come ha detto il Ministro della giustizia, abbiamo necessità di sapere la verità. Quello che è avvenuto, se fosse nei termini in cui appare dai giornali, è certamente un problema di vitalità del nostro Paese

ideale che mi portava a ritenere che la Costituzione dice qualcosa che rappresenta il popolo italiano. Quella era la filosofia della Commissione dei 75. La filosofia della Costituzione sui detenuti ha un valore enorme. Dobbiamo renderci conto che i detenuti vivono in una situazione di ristrettezza,

forse non avendo nemmeno gli strumenti per poterli compiere legittimamente.

nella forza di coloro che non hanno voglia di chiudere le persone in carcere e buttar via la chiave; non è questo il modo di essere del nostro Paese.

sconcertante mette anche in evidenza che, all'interno delle carceri, da troppo tempo vi sono condizioni, sia per chi vi lavora, sia per chi è detenuto, non all'altezza di quelli che dovrebbero essere gli *standard* di un Paese come il nostro.

chiedere un impegno al Governo, ciò è chiaramente per rendere anche possibile lavorare all'interno delle carceri in maniera sicura e certamente giusta. Dopodiché, tra le guardie e i ladri, noi non abbiamo dubbi: noi stiamo sempre con le guardie. Bisogna garantire a chi viene carcerato la sicurezza, ma bisogna garantire a chi svolge il proprio dovere in uniforme di non subire anche condizionamenti rispetto a un sistema che vuole mettere i numeri sopra le guardie carceraria e la Polizia penitenziaria, come se fossero loro i carcerati. Signor Presidente, ci siamo posti anche un quesito, una domanda su una cosa molto curiosa. Da tempo, infatti, insistiamo nelle Aule del Parlamento affinché il Governo capisca che, inserire all'interno di luoghi delicati, dove possono esserci maltrattamenti, sistemi di controllo con le telecamere è un'opportunità per garantire legalità.

di maltrattamenti. Tuttavia, se lo dice la Lega, non va bene; se lo dice Salvini, si deve dire l'opposto. Quanto accaduto ci deve far riflettere quindi sotto molti punti di vista, anche sul piano della tutela di chi è in condizioni di essere offeso senza potersi difendere.

sia per contenere, sia per tutelare chi vi lavora e chi vi viene recluso. Su questo abbiamo bisogno che il Ministro venga in Aula a riferire, dandoci certezza sul fatto che il Governo non sta sottovalutando la situazione, anche l'onorabilità di un corpo come quello della Polizia penitenziaria, che per nulla può venire macchiato dal comportamento di singoli individui.

In quei giorni però, a differenza di tanti colleghi che adesso parlano in questa sede, io sono andato lì con altri miei colleghi a portare vicinanza e solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria, per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono nelle carceri, in un posto difficile come il carcere di Santa Maria Capua Vetere. *(Applausi).* Sono entrato anche nei bracci nei bracci del carcere, ho parlato con i detenuti e negli occhi di alcuni si percepiva la paura di parlare. A tal riguardo auspichiamo che le indagini facciano il loro corso. Questo è il settore giusto. sono intervenute delle immagini fortissime, che tutti abbiamo visto, e anche dei messaggi scritti da alcuni agenti che fanno sembrare che l'azione sia stata premeditata. Questo non va bene, perciò rilanciamo la richiesta affinché la ministra Cartabia venga a riferire in Aula per fare chiarezza, affinché la garanzia della custodia e la funzione rieducativa della pena, sancite dalla nostra Carta

Il ministro D'Incà era presente quando è stato sottoposto il problema; segnaleremo queste ulteriori richieste che vengono all'unanimità da tutti

Signor Presidente, una serie di terrificanti incendi ha attraversato la Sicilia negli ultimi giorni. Nessuna Provincia è stata risparmiata dal fuoco che ha divorato ettari di macchia, boschi e campi coltivati, con la perdita dei raccolti; centinaia di cittadini sono stati evacuati dalle loro case, poste sotto assedio dalle fiamme che hanno interessato alcune aree protette, facendo strage di fauna selvatica e biodiversità. Sono state colpite troppe aziende agricole, con immobili, attrezzature e capi di bestiame; famiglie di agricoltori hanno perso tutto: il lavoro e le speranze di una vita. In alcuni casi gli incendi hanno lambito le aree archeologiche, mettendo a rischio il patrimonio culturale siciliano. Si tratta di un disastro ambientale, economico e umano. Cittadini e agricoltori hanno dovuto difendere personalmente casa e beni, combattendo le fiamme accanto alle donne e agli uomini della Protezione civile, ai Vigili del fuoco e al Corpo forestale, cui va la riconoscenza del MoVimento 5 Stelle per lo spirito di sacrificio con il quale affrontano questa emergenza Ad impressionare quest'anno sono le proporzioni del fenomeno, che tuttavia non rappresenta alcuna novità. A nulla è valso l'appello che nei mesi scorsi ho rivolto alle autorità regionali, chiedendo di potenziare e accelerare l'attività di prevenzione. La negligenza della politica regionale è evidente: basti guardare al Corpo forestale regionale, che negli anni è stato penalizzato nella capacità operativa, con mezzi obsoleti, carenza di personale, pochissimi ispettori, guardie forestali in numero esiguo e spesso in età avanzata. Il tutto nell'ambito di un piano antincendio regionale che di fatto risulta tardivo e inefficace. La Sicilia ha una legge regionale che tutela il patrimonio vegetale, il secondo più basso indice di copertura forestale a livello nazionale, ma è tra le prime Regioni per numero ed estensione degli incendi: mi chiedo perché. È possibile che ci siano interessi speculativi legati ai servizi antincendio o al mercato fondiario? Nella speranza che la magistratura trovi elementi utili a rispondere a queste domande, bisogna intervenire valutando, valutando, ad esempio, l'utilizzo dei droni Predator in dotazione all'aeronautica militare che, attraverso il telerilevamento con camere termiche, possono vigilare sui territori, individuando precocemente i focolai in modo più efficace ed economico rispetto al dispiegamento di migliaia di militari, come richiesto dal presidente Musumeci. Allo stesso modo occorre inasprire le pene per i criminali che bruciano il nostro futuro, equiparando l'incendio delle aree rurali a quelle boschive. Domani i cittadini della Provincia di Enna scenderanno in piazza spontaneamente chiedendo risposte alle istituzioni. L'incapacità della Regione Siciliana di gestire l'emergenza incendi è sotto gli occhi di tutti e allora, se la Sicilia brucia, lo Stato ha il dovere di intervenire a tutela dell'ambiente e dell'incolumità dei cittadini.

finendo di fatto nel tessuto urbano di una città di 100.000 abitanti. Tale impianto, come tanti similari in Italia, è utilizzato come co-inceneritore di rifiuti pretrattati CSS e ciò desta forte preoccupazione. A febbraio 2019, per conoscere i possibili effetti degli inquinanti emessi, pur monitorati a camino e nei limiti di legge, è stato siglato un protocollo d'intesa tra Comune, ASL, comitato ISDE, ordine dei medici, scuole primarie e associazioni ambientaliste per un biomonitoraggio finanziato dalla ASL. La proposta fu lanciata dal Forum salute ambiente, portata nelle istituzioni dai consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle e, grazie alla pressione di tanti cittadini, attuata dal sindaco.

Il 25 giugno scorso, il dottor Di Ciaula ha pubblicato i risultati dello studio sulla prestigiosa rivista Exposure and Health. I bambini che vivono e frequentano la scuola nell'area esposta alle emissioni del cementificio mostrano un bioaccumulo cronico di metalli tossici, quali nichel, cadmio, mercurio e arsenico. Questi si correlano indicando una fonte comune. L'articolo conclude che i cementifici situati in aree urbane sembrano dannosi e che quindi sono necessarie politiche di prevenzione primaria per proteggere la salute dei bambini, delocalizzazione, norme più restrittive per l'uso dei combustibili fossili, limitazione di rifiuti ricchi di metalli pesanti, educazione sanitaria. Questo Questo studio impone ora la massima attenzione, nazionale e non solo, sia sul fronte sanitario, per approfondire e valutare l'effettivo rischio sui residenti nei dintorni dei cementifici, sia su quello ambientale e socio-economico, al fine di eliminare la causa, se è pericolosa. Bruciare i rifiuti, così come tombarli, è un tragico errore e ora sappiamo che potrebbe essere anche pericoloso, ancor più per i bambini.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi prenderò la libertà di intervenire, oltre che da senatrice, anche da mamma, perché è inaccettabile che in un Paese civile si possa morire mentre si prende il sole o si gioca in un parco. Mercoledì 23 giugno, intorno alle 12,30, un giovane, residente poco lontano dal mio Comune e spinto da un impulso di far del male, ha scelto a caso una vittima, una giovane donna che stava prendendo il sole lungo il fiume Piave. L'ha aggredita alle spalle e l'ha trafitta con varie coltellate prima di tagliarle un orecchio, che si è portato via come un trofeo. Volevo qualcosa che me la ricordasse, ha dichiarato il giovane in Questura. Egli era seguito dal centro di igiene mentale della zona, ma sembra non assumesse i farmaci. Il 13 giugno scorso due bambini, due figli, due nipoti, persi in un attimo per la follia di un altro soggetto, che è stato letteralmente abbandonato dalle istituzioni. Lo voglio ricordare di nuovo qui, perché i fatti di cronaca si dimenticano velocemente e ciò non dovrebbe accadere. La dura e cruda realtà è che dobbiamo ricordare che due bambini di cinque e dieci anni non ci sono più. È un dolore lacerante, che grida giustizia. Basta nascondersi dietro un dito. Sono troppi i casi di soggetti psichiatrici, di infermità di mente, che sfociano in omicidio. Molti di questi casi, poi, erano praticamente annunciati nella loro evidente prevedibilità. Le ultime disgrazie accadute ci mettono nuovamente di fronte a come la legge Basaglia sia rimasta a metà del guado per la prematura morte di chi l'ha voluta e i suoi successori non sono stati in grado di comprenderne la visione. È così rimasta incompiuta una riforma che voleva portare alla luce le ingiustizie commesse all'interno dei manicomi e che ora condanna i pazienti e le loro famiglie a uno stato di abbandono. Il sistema italiano non è stato in grado di mettere in piedi il segmento della cura. Le famiglie sono state lasciate colpevolmente sole, riducendo il tutto a mere classificazioni dottrinali e a prescrizioni farmacologiche. Mi spiegate con quali strumenti possa chiedere aiuto una persona che sta male? Come fa? Perché i familiari non possono agire per il proprio figlio? Al massimo vengono dati sette giorni di trattamento Questo è un colpevole abbandono delle istituzioni, un sistema che dimentica le necessità di troppe famiglie in queste condizioni. Questo assordante silenzio, il dire «non è colpa nostra» non basta per lavare la nostra coscienza da responsabilità del genere, da queste morti, come da tutte quelle avvenute senza che noi ci scandalizzassimo, se non per un breve periodo, magari davanti ai riflettori, per poi lasciare tutto come sta, coerenti con il nostro malcostume tipico. Basta. Con la senatrice Marino lo stiamo dicendo da inizio legislatura: le persone hanno diritto alla cura, le famiglie hanno diritto ad essere aiutate e lo Stato deve smettere di far finta di nulla. *(Applausi)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in Aula per una situazione abbastanza preoccupante e per le preoccupazioni manifestate soprattutto da molti docenti circa le dichiarazioni del professor Miozzo, che che è il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico. Si tratta di dichiarazioni che portano addirittura a presagire misure atte a obbligare i docenti a effettuare le vaccinazioni per la didattica in presenza, cosa che assolutamente, allo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche, è inaccettabile. È inaccettabile perché è stato lo stesso Comitato tecnico-scientifico a cambiare versione sui vaccini

poi sospeso precauzionalmente in tutta Italia, poi autorizzato per tutti i maggiorenni, poi raccomandato agli *over* sessanta con *open day* accessibili a tutti, poi *stop* per chi ha meno di sessant'anni e seconda dose con Pfizer o Moderna, poi libertà di scelta per la seconda dose, con il consenso informato. Insomma, signori miei, se questo Comitato tecnico-scientifico non sa dove deve andare, come può permettersi di obbligare chicchessia ad effettuare una vaccinazione sperimentale in un Paese in cui si impone chiaramente il consenso informato? Il cittadino ha diritto di scegliere a quale trattamento sanitario assoggettarsi. Tutto questo è assolutamente inaccettabile. Per tenere le scuole aperte basta semplicemente ridurre il numero degli alunni per classe, provvedimento che nessuno vuole mettere in campo. Esistono tanti istituti scolastici dismessi, abbandonati, che possono essere utilizzati o ripristinati per poter creare classi aggiuntive, per ridurre la possibilità di contagio e consentire a tutti la frequenza in presenza. Quindi si accetti, una volta per sempre, di aumentare la spesa corrente sull'istruzione, per garantire a tutti i cittadini di istruirsi in sicurezza e nella libertà di scelta

alle quali risponderanno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'università e della ricerca. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

richiamo quanto accaduto, ad esempio, con il tentativo croato di copiarci la denominazione "Prosecco", a me caro anche per ragioni regionali. Ciò dimostra quanto l'agricoltura italiana sia assolutamente sotto tiro.

in Europa del 10 per cento, che però in Italia si traduce in un taglio addirittura del 15 per cento, con una serie di impegni molto più stringenti rispetto a prima e addirittura con meno risorse. Ricordo a tutti che il taglio del 15 per cento in Italia vale circa

se lei abbia fatto una valutazione di impatto sulle nuove norme e le nuove modalità della PAC, e come intende rendere il Parlamento edotto e partecipe di quelle scelte che il Piano strategico dovrà fare di qui a breve per dare contezza della nuova PAC.

perché, se vogliamo proteggere - come vogliamo - la distintività delle nostre produzioni agroalimentari, dobbiamo farlo concentrando le risorse. Vado, pertanto, al punto della quantità di risorse. È vero che c'è un taglio di 6,2 miliardi nel settennato delle risorse sulla PAC per il nostro Paese, ma è anche vero che nel quadro finanziario pluriennale europeo l'aver individuato 750 miliardi per il Next generation EU ha fatto sì che - da un lato - abbiamo perso quelle risorse parcellizzate sulla PAC e - dall'altro - abbiamo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 7,9 miliardi

per fornire ai cittadini cibo in quantità e sicurezza. Lo scopo primario della PAC è sostenere gli agricoltori nella produzione. Con 6,2 miliardi in meno

grandissimo plauso da tante parti politiche, prevede una perdita di produttività dei terreni di circa il 7 per cento. E come se non bastasse, la stessa

all'agricoltore il prezzo dei nostri cambiamenti. Se per qualcuno l'agricoltore è una vacca da mungere, ricordo a tutti che a quella vacca prima bisogna dare da mangiare.

a parte i problemi di riduzione del reddito delle nostre aziende agricole per via di una PAC che in ogni settennio vede ridurre i trasferimenti verso gli agricoltori italiani e, in particolare, verso quelli del Mezzogiorno, l'agricoltura italiana soffre - penso, in particolare, ai cerealicoltori del Sud in Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia - perché deve anche affrontare la concorrenza internazionale spietata

grazie a un'Unione europea compiacente con limiti su contaminanti più elevati addirittura dell'Africa, diventa il porto di ultima istanza per tali navi. Ieri è approdata in Italia una nave carica di grano duro canadese, una *bulk carrier*, denominata Sumatra, battente bandiera portoghese, che è arrivata a Ravenna dopo essere stata respinta dalle autorità dell'Algeria nel porto di Annaba per motivi sanitari, come ci riferiscono fonti giornalistiche straniere. Al suo interno sono stati trovati insetti, un odore sgradevole, infiltrazioni d'acqua e sicuramente delle muffe. La nave, dopo circa un mese, ha ripreso il mare il 30 giugno e, dopo un breve rifornimento presso il sito di Sarroch in Sardegna, si è diretta verso Ravenna. Secondo una dichiarazione dell'ufficio di presidenza del porto di Annaba, la spedizione è stata respinta perché non conforme agli *standard* qualitativi concordati tra gli importatori africani e il fornitore Richardson. Dunque presso un porto italiano è arrivata una nave fortemente sospettata di trasportare un carico di grano deteriorato e ammuffito. Ora, considerato che ci sono tutti gli elementi per intervenire e controllare detta nave prima che inizino le procedure di scarico; considerato che probabilmente qualcuno destinerà quella nave anche ad uso zootecnico, se non dovesse essere adeguata per uso alimentare, io le chiedo di intervenire e di portare i livelli

sollevate afferiscono al settore cerealicolo, all'importazione di grano nei porti italiani e in particolare all'arrivo presso il porto di Ravenna di una motonave con un carico di grano che si presume, in modo abbastanza evidente, avariato. Trattasi di materie che concernono la salubrità e gli aspetti igienico-sanitari del grano trasportato nelle stive delle navi, soggetto ad attacchi di parassiti e altre alterazioni a causa dei tempi lunghi di stivaggio. Tali aspetti rientrano nelle competenze dei Posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute preposti ad effettuare le verifiche sia sugli alimenti che sui mangimi. A tal riguardo informo che abbiamo prontamente contattato gli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) di Ravenna, i quali ci hanno riferito che la nave MV Sumatra è al momento all'ormeggio in rada presso il porto di Ravenna. Gli uffici sanitari sono in stretto contatto con il responsabile antifrode della dogana per un aggiornamento continuo. La situazione allo stato pare sotto controllo e non c'è ovviamente l'autorizzazione allo sbarco. In linea generale, evidenzio che sugli alimenti di origine vegetale, la Commissione europea, sulla base delle valutazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), dispone specifiche percentuali di controllo sulle partite a rischio per determinati pericoli, in rapporto al Paese di provenienza. Anche il nostro Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione le modalità di conservazione o l'effettuazione di eventuali trattamenti per le granaglie stoccate nei silos; vengono inoltre esaminati i documenti di accompagnamento e di rintracciabilità della merce; il rispetto dei parametri analitici di riferimento; l'eventuale presenza di sostanze attive ad azione fitosanitaria impiegate nel campo e in post raccolta; il processo di trasformazione dei prodotti derivati dalle farine e dalle semole; il rispetto delle norme di etichettatura, della conformità e veridicità delle indicazioni obbligatorie e facoltative, con particolare riguardo all'origine geografica riportata sui dispositivi di etichettatura e sui documenti commerciali. Per aumentare l'efficacia dei controlli all'importazione, I'ICQRF ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto al fine di disporre di dati e di informazioni sui trasporti marittimi di prodotti agroalimentari e di mezzi tecnici di produzione agricola, monitorare le introduzioni sul territorio nazionale, effettuare ispezioni congiunte al personale delle medesime capitanerie capitanerie ed avere un accesso facilitato sulle navi e ai *containers* trasportati. Inoltre, per contrastare in modo più incisivo l'eventuale illecita importazione di prodotti agroalimentari sul territorio nazionale, da anni è stato instaurato un rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per poter monitorare i flussi in entrata di alimenti e materie prime alimentari provenienti da Paesi extra UE e impedire l'ingresso di prodotti privi della documentazione di tracciabilità, ovvero non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi, stabiliti dalle norme di settore. Grazie all'acquisizione della strumentazione tecnico-scientifica all'avanguardia, è stata ulteriormente potenziata l'attività analitica di controllo di laboratorio dell'ICQRF, consentendo rapide ed efficaci strategie di *screening* volte a rilevare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi di metaboliti, ivi compreso il glifosato, nonché di eventuali adulteranti. Questo collaudato sistema di controlli garantirà, anche nei confronti del caso specifico segnalato all'interrogante, che vengano effettuate tutte le verifiche necessarie sulla tracciabilità, la qualità e l'effettiva destinazione dei grani importati, al fine di impedire che gli stessi siano illecitamente commercializzati nel nostro Paese, nel caso in cui venissero accertate difformità del prodotto rispetto a

confido nell'impegno che vorrà dedicare alla questione cerealicola per l'Italia. Le voglio sintetizzare che il

di terza categoria "western amber durum", proveniente da Vancouver, abbia una sua tipologia merceologica e tossicologica. All'estero (negli Stati Uniti, in Canada e in Australia), la qualità tossicologica viene valutata in modo rigoroso. So bene che il Ministero sta affrontando questo tema con la Commissione unica nazionale, che dovrebbe armonizzare i prezzi italiani con quelli internazionali. Sin da quando c'era il ministro Martina, la stessa Ismea ha sempre dichiarato che questa armonizzazione in Italia non c'era, lasciando spazio a operazioni di

qualitativo e quantitativo, per una giusta previsione dei prezzi in Italia e per un'armonizzazione con i prezzi internazionali. Signor Ministro, premesso che nelle ultime settimane abbiamo assistito a un crollo del prezzo dei cereali di provenienza estera, che sta causando il crollo del mercato italiano, la Commissione unica nazionale sul grano dovrebbe costituire un osservatorio stabile sui prezzi, contribuendo a criteri di maggiore trasparenza. Esiste però un evidente sperequazione tra territori e filiere e sedi delle commissioni uniche nazionali, che richiede una maggiore presenza del Meridione, in quanto rappresenta un importante apporto alla produzione nazionale. Il tema della concorrenza sleale sul grano attiene anche alle questioni sanitarie legate all'importazione, al trasporto e all'immagazzinamento dei grani di provenienza estera, il cui controllo deve tutelare maggiormente la sicurezza dei consumatori italiani. Il prezzo più alto del grano italiano è proprio conseguente a procedure e oneri ulteriori che gravano sui produttori italiani, in quanto soggetti a maggiori protocolli di sicurezza e di controllo per la gestione dell'intero ciclo produttivo. Allo stesso modo, tutti gli altri prodotti alimentari italiani sono soggetti a procedure di produzione e cessione sul mercato, che comportano oneri ulteriori rispetto ai prodotti di provenienza estera, sempre a tutela della qualità del prodotto italiano che va sulle tavole dei consumatori. chiediamo di sapere: cosa intenda fare il Ministro per tutelare il reddito dei produttori agricoli italiani, che garantiscono sicurezza alimentare del grano e degli altri prodotti alimentari, ma sono soggetti a maggiori oneri di produzione; considerata la stagione di siccità nella quale siamo e le diverse calamità naturali verificatesi, soprattutto nel Sud Italia, quali misure straordinarie siano previste per ristorare gli agricoltori, che a fine anno porteranno un conto salatissimo, e in che modo si possa al contempo intervenire sulla questione delle assicurazioni agricole; a che punto sia la creazione di un marchio che certifichi e valorizzi la totale italianità al 100 per cento di un prodotto alimentare italiano.

dipende da diversi fattori e, per sostenere il comparto, occorre agire su diversi fronti, come la trasparenza dei prezzi, la competitività del settore e l'integrazione di filiera. In tale direzione, per una più limpida e condivisa quotazione del grano duro, stiamo dando avvio alla CUN, la Commissione unica nazionale sperimentale, per la quale è stato recentemente definito il regolamento di funzionamento tra la parte venditrice, cioè le associazioni di parte agricola, e la parte acquirente, Italmopa. Siamo quindi in procinto di una fase storica nella formazione del prezzo del grano duro che consentirà anche di riequilibrare i rapporti di filiera. Inoltre, per garantire un aiuto al reddito degli agricoltori, dal 2016 è attivo il "Fondo grano duro", rifinanziato da ultimo con la legge di bilancio del 2020 e attuato con il decreto 20 maggio 2020, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro. Tale fondo prevede l'erogazione di un contributo pari a 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno-inverno dell'annualità precedente in favore di imprese agricole che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, contratti di filiera di durata almeno triennale. I contratti di filiera sono infatti uno dei principali mezzi di sostegno alle politiche agro-industriali gestiti dall'amministrazione e strumento di finanziamento che si adatta bene a un tema di sviluppo economico del settore dei cereali e in particolare del grano duro, per migliorare l'integrazione tra i diversi operatori della filiera. Sui contratti di filiera il fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede 1,2 miliardi Riguardo alla valorizzazione dell'italianità del prodotto, unita a una corretta informazione al consumatore, ricordo che è già stata introdotta l'indicazione d'origine in etichetta del grano duro per pasta di semola di grano duro, con l'intento di rendere evidente anche la provenienza della materia prima, oltre che quella del prodotto finito. Per quanto concerne, infine, le misure per la copertura dei rischi delle colture cerealicole nazionali, siamo riusciti a ottenere nella PAC l'aumento dall'1 al 3 per cento del prelievo sul primo pilastro per la gestione del rischio. Rilevo che gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative agevolate da contributi europei, cofinanziati con risorse nazionali fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta. Inoltre, per il settore del frumento per il settore del frumento è attiva da alcuni anni una misura di aiuto sulla spesa assicurativa agevolata con risorse nazionali, che consente la sottoscrizione di polizze a copertura dei ricavi, comprese, quindi, le oscillazioni di prezzo come quella segnalata. Non dobbiamo comunque dimenticare che le assicurazioni agricole agevolate, cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 2,1 miliardi di euro per il periodo 2015-2022, rappresentano il principale strumento di intervento messo in campo dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito subite dalle imprese agricole in caso di avversità atmosferiche. Rilevo inoltre che l'attività di comunicazione avviata nell'ambito del programma di sviluppo rurale nazionale, finalizzata tra l'altro ad ampliare la conoscenza degli strumenti a disposizione, ha portato a un lieve, ma costante aumento della sottoscrizione di polizze agevolate. Per la prossima programmazione dei fondi comunitari relativi allo sviluppo rurale stiamo infine approntando un nuovo strumento di intervento *ex ante* sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale proprio grazie alla possibilità di aumentare il prelievo. Con le risorse del primo pilastro PAC il 30 per cento sarà a carico dell'agricoltore e il 70 per cento con le risorse del FGASR del secondo pilastro. Questa possibilità, che è già stata richiesta e ottenuta dall'Italia grazie all'impegno del Governo e ai nostri parlamentari europei, consentirà di ampliare notevolmente la diffusione degli strumenti di gestione dei rischi a territori e settori come quelli segnalati ad oggi non adeguatamente coperti. ringrazio il ministro Patuanelli per la puntuale risposta a un quesito che, per la sua ampiezza e la miriade di questioni ad esso collegate, non era di semplice argomentazione. La questione della produzione e approvvigionamenti agricoli espone l'Italia alla volatilità dei prezzi questo lo ha spiegato bene - quindi, posso ritenermi soddisfatta. Vorrei utilizzare il tempo per pungolare l'Esecutivo, quindi, lei, Ministro. Ecco perché vorrei ritornare ancora una volta sul disagio che vivono i nostri impegni agricoli a causa dei fenomeni climatici. Penso alle gelate, ma anche alle improvvise piogge torrenziali e grandinate. Cito solo un episodio episodio come esempio, ovvero quanto accaduto lo scorso 12 giugno in Calabria, dove la grandine da *record* ha distrutto il raccolto di frutta, in particolare pesche e ortaggi. Dinanzi a fenomeni del genere, sempre più frequenti proprio a causa dei cambiamenti climatici, uniti alla presenza della fauna selvatica - di cui discuteremo prossimamente - che ci ha visti stamattina insieme sullo stesso palco per la manifestazione di Coldiretti, ma che avrebbe dovuto vederci insieme anche in quest'Aula stamattina, come richiesto da Forza Italia e da tutto il centrodestra per approvare in Assemblea quanto già fatto in Commissione agricoltura, c'è necessità di provvedimenti incisivi e di certezza del sostegno. Anche e soprattutto questo è un modo di sostenere il reddito dei nostri imprenditori, tutelando le nostre aziende produttrici di qualità nonché dell'intero circuito, a partire dalle forti braccia di uomini e donne che ogni giorno lavorano i nostri campi. Non lasciamo soli i nostri agricoltori, altrimenti a chi verrà affidato il compito di curare il nostro bellissimo patrimonio naturale, contrastandone l'abbandono?

*(L-SP-PSd'Az)*. Signor Ministro, il falso *made in Italy,* secondo le recenti stime, ha ormai superato abbondantemente i 100 miliardi di euro l'anno. Teniamo conto che l'*italian sounding* è cresciuto del 70 per cento negli ultimi dieci anni. Questo fenomeno che falsifica la realtà del *made in Italy* con l'uso di parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette inganna il consumatore, evocando l'origine italiana di alimenti che sono privi di qualsiasi legame col nostro territorio. Il tema di oggi è quello del vino, signor Ministro, e nello specifico della difesa del nostro Prosecco. Il fatturato delle aziende italiane che producono vino ha superato gli 11 miliardi di euro, le aziende che vinificano sono oltre 40.000 e impiegano oltre 35.000 addetti.

Signor Ministro, la nuova battaglia in cui siamo chiamati in difesa sta coinvolgendo il Prosecco ed è iniziata con la presentazione alla Commissione europea da parte della Croazia della denominazione di registrazione della menzione tradizionale "Prosek" per un vino bianco fermo prodotto sul territorio croato. Già nel 2013 Zagabria aveva provato a registrare la stessa denominazione per un passito e l'avrebbe denominato anche "Prosek"*.* Allora, la Commissione europea aveva respinto la domanda, perché il marchio di denominazione di origine protetta era già stato assegnato al Prosecco italiano. Questa volta la preoccupazione dei produttori è legittima, perché la domanda potrebbe venire accettata almeno per quanto riguarda la pubblicazione sulla Gazzetta dell'Unione europea, un primo passo che non significherebbe il via libera a questa vergognosa domanda, ma comunque un avvio di un periodo di due mesi in cui gli enti pubblici e privati potranno presentare le loro osservazioni ed i motivi per cui ritengono che non debba essere accolta. Vogliamo da subito sentire da lei che il Governo italiano e il Ministero si impegnano ad una formale e netta posizione contro questa richiesta che è tra l'allucinante e il catastrofico. Il Prosecco è solo italiano, così come sono italiane le colline di Conegliano e di Valdobbiadene dove si coltivano i vitigni. Queste terre - non dimentichiamocelo - sono iscritte nella lista UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Questa iscrizione non ha un valore simbolico, ma significa riconoscere e decretare

di proteggere le nostre produzioni DOP, IGP e tutte le nostre produzioni distintive in generale. Prosecco è una frazione del Comune di Trieste, quindi può immaginare se non sarò a difesa del Prosecco, della sua eccellenza e della sua qualità. Mi preme innanzitutto rassicurare sul fatto che ci siamo già attivati presso la Commissione europea opponendoci in modo formale all'accoglimento della domanda di registrazione di menzione tradizionale (MT) "Prosek" presentata della Croazia, nonché alla relativa procedura di procedura di pubblicazione, quindi è già un atto. In occasione del Comitato di gestione OCM del 29 giugno scorso abbiamo infatti rappresentato la nostra ferma contrarietà all'accoglimento della richiesta in questione, in quanto la menzione corrisponde, in traduzione, al nome della DOC "Prosecco" e delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco", in netto contrasto con la normativa europea di riferimento diretta a proteggere i prodotti iscritti nel registro delle DOP della Commissione europea. A supporto della nostra posizione, abbiamo altresì evidenziato che sin dai primi negoziati per l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea era stata avanzata dalla stessa Croazia una medesima richiesta che, su nostra opposizione, non fu accolta né successivamente recepita, come ricordava il senatore Bergesio, nei regolamenti e nelle decisioni relative al Trattato di adesione, né iscritta nell'apposito registro della Commissione. Assicuro quindi che è ferma intenzione del Governo continuare a seguire con estrema attenzione la questione rappresentata al fine di garantire alle nostre produzioni la tutela che meritano e per contrastare tutti i possibili attentati - è giusto chiamarli così - alle nostre prestigiose DOP e IGP, non ultime le usurpazioni di carattere commerciale che vengono perpetrate sui siti Internet. Purtroppo è ancora fresco il

quindi noi dobbiamo prepararci a una guerra che è già in atto, perché già nel 2013 c'era stato un tentativo di attaccare queste eccellenze del *made in Italy*;

Particolare attenzione va rivolta al Prosecco, che è sicuramente una colonna portante dell'agricoltura italiana. Io vengo dal Veneto, dalla provincia di Treviso, così come lei è di Trieste e la sento molto vicino in questa situazione. tutta l'agricoltura italiana è sotto attacco, l'*italian sounding* ci costa oltre 100 miliardi di euro, quindi uniamoci tutti a difesa della nostra agricoltura.

Presidente, signora Ministra, noi parliamo delle borse di specializzazione dei giovani medici. Nell'ultimo anno, come Governo e Parlamento, abbiamo aumentato i posti messi a disposizione, tuttavia l'attuale sistema delle scuole di specializzazione in medicina sembra non prevedere di fatto la formazione di un numero sufficiente di specialisti per i prossimi anni, in una contingenza resa ancora più drammatica dal *post* Covid e alla luce dei tanti pensionamenti che ci saranno nei prossimi cinque-dieci anni. Ogni anno 1.500 laureati in medicina decidono di trasferirsi all'estero, collocando l'Italia al primo posto in Europa per migrazione dei giovani medici. In più, il personale medico in Italia è il più anziano d'Europa. La formazione dei giovani medici e, a mio avviso, anche quella dei medici di medicina generale, che dovrebbe essere equiparata alle scuole di specializzazione, acquisisce un rilievo importantissimo per lo sviluppo del nostro Paese nei prossimi mesi. Alla luce della direzione assunta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli investimenti in strutture e tecnologie (dalla digitalizzazione alla telemedicina, all'intelligenza artificiale) dovranno essere necessariamente accompagnati anche da una forte valorizzazione delle risorse umane. chiedo, quindi, quali sono i suoi orientamenti in proposito, se non ritenga opportuno abbattere l'imbuto formativo dei giovani medici nell'accesso alle specializzazioni, prevedendo un numero sufficiente di borse per i prossimi anni, anche allargando le reti formative, per esempio alla rete dei presidi sanitari territoriali. La medicina territoriale, infatti, è il tema principale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per evitare ospedali pollaio, con il sovraffollamento di personale in formazione. Le chiedo, infine, se non ritenga necessario riformare le modalità di accesso e di permanenza presso le scuole di specializzazione, al fine di rendere maggiormente convergenti le aspirazioni e i desideri di specializzazione dei giovani e delle giovani medico con le borse effettivamente disponibili, alle quali hanno accesso.

la determinazione del quantitativo di borse di specializzazione medica consegue a un articolato e complesso processo, che origina dalla individuazione del fabbisogno di medici specialistici sul territorio nazionale da parte del Ministero della salute e prosegue poi con il reperimento delle risorse necessarie,

Su questo punto voglio dire che è già stato fatto molto e si farà ancora di più al fine di ampliare la rete formativa, grazie al lavoro che sta svolgendo oggi, e che ha svolto anche negli anni passati, l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria a cui partecipano anche rappresentanti del MUR e della salute e che ha espressamente rivolto delle raccomandazioni agli atenei, invitandoli ad ampliare le reti formative soprattutto per quelle scuole dove è constatata una necessità a causa della esiguità delle stesse. Con riferimento, invece, al tema del numero delle borse di specializzazione, va detto che in questi anni, anche grazie all'attenzione del Parlamento, si è assistito a un *trend* in costante crescita.

stiamo lavorando in questi anni sul cosiddetto imbuto formativo, ma riteniamo che debbano essere ulteriormente aumentati i posti per andare incontro a un periodo di fabbisogno decisamente aumentato. aumentato. Tale aumento, che viene programmato e del quale stiamo discutendo insieme al Ministero della salute e al MEF, spero che si verifichi già a partire da quest'anno, dalla prossima tornata. Il compito importante del mio Ministero è poi quello di garantire una giusta articolazione dell'offerta formativa. Voglio anche comunicare che dell'università e della ricerca promuoverà anche un'armonia fra il fabbisogno e le leve motivazionali al fine di assicurare la continuità formativa dei nostri medici.

virtuosa tra Governo e Parlamento faremo tutti la nostra parte. Mi piace molto quello che ha detto al termine del suo intervento in merito al fatto che il suo Ministero deve assicurare l'articolazione dell'offerta formativa e l'armonia tra fabbisogno e motivazione. A tale proposito le dico che noi prima di essere parlamentari siamo cittadini e abbiamo visto

Li abbiamo messi in prima linea, dagli ospedali Covid, alle USCA, agli *hub* vaccinali. Sappiamo tutti il lavoro che stanno svolgendo, un lavoro anche di organizzazione, di prenotazione dei vaccini, di accompagnamento psicologico alla cittadinanza, un lavoro in squadra con gli altri protagonisti di queste vaccinazioni che sono gli infermieri e i volontari. Penso quindi che dovremmo trovare un modo - ripeto - per valorizzare l'impegno grandissimo dei giovani medici e dei medici in generale. La politica non solo deve ringraziarli, ma anche valorizzare il lavoro

Signora Presidente, signora Ministro, al centro della nostra interrogazione c'è il diritto allo studio, un tema politico rilevantissimo in particolare in questa fase di crisi così dura, che mortifica le aspettative e le speranze di tanti che sono più deboli e più colpiti dagli effetti della pandemia, in particolare i più giovani, perché poter studiare significa potersi emancipare. Sappiamo che la crisi rischia di impedire a moltissime ragazze e ragazzi di continuare a studiare e quindi di rinunciare alla cosa più importante che hanno, che abbiamo, che è il nostro progetto di vita. Se non interverremo - ma noi dovremo intervenire - la nostra società sarà più debole. Investire nel diritto allo studio significa invece dare forza a energie vitali, liberare energie che sono fondamentali non solo per i destini individuali, ma collettivi, per il nostro Paese, per il suo ruolo nel mondo. In un Paese come il nostro, in cui studiare è già difficile, abbiamo un numero troppo basso, tra i più bassi in Europa, di immatricolati, di laureati e di ricercatori; chi chi viene da un istituto tecnico professionale deve superare una barriera a volte invalicabile per poter accedere all'università e continuare a studiare e a laurearsi sono nella quasi totalità i figli di chi è già laureato. Ecco, se dopo la pandemia dobbiamo costruire un nuovo modello di sviluppo, al centro deve esserci il diritto allo studio. Con grande forza politica abbiamo in questi anni fatto conquiste importanti, grazie anche alle nostre battaglie, che voglio ricordare: quella sulla *no tax area* e quella capace di raddoppiare i fondi statali per le borse di studio. Tuttavia il nostro è un sistema ancora troppo fragile, con troppe differenze tra Regione e Regione, con il rischio di desertificazione di interi territori; è un sistema con una tassazione troppo alta. Per questo, signor Presidente, abbiamo voluto, su nostra proposta, che il Senato portasse avanti un'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca. Per questo, signora Ministro, oggi le chiediamo di esercitare con urgenza la delega sui livelli essenziali delle prestazioni, per riconoscere - come scritto in Costituzione - a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti di istruzione. Signor Presidente, i senatori hanno toccato un tema molto complesso, che riassumo molto brevemente. L'attuazione delle norme di legge in tema di diritto allo studio non è ancora completata.

fu presentato alla Conferenza Stato-Regioni nel 2013, ma non raggiunse l'intesa. In quella occasione le Regioni espressero la volontà di poter operare una ricognizione delle prestazioni da esse effettivamente offerte prima di cristallizzarle nei LEP. Questa sospensione del processo di individuazione dei LEP non ha impedito, in ogni caso, l'emanazione di un altro decreto interministeriale, il n. 798 del 2017, con il quale si è potuto dare attuazione a una parte significativa del citato decreto legislativo n. 68. Con tale decreto il Ministero ha provveduto infatti alla definizione dei fabbisogni finanziari delle Regioni, nonché alla definizione dei criteri e modalità di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS). Sulla base di questo decreto si è proceduto, nel triennio 2017-2019, all'assegnazione delle risorse del FIS in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni, prevedendo anche meccanismi premiali per le Regioni che avevano investito maggiori risorse sul diritto allo studio. Inoltre, al termine del triennio, in accordo con le Regioni, si è ritenuto di intervenire sul decreto con alcuni correttivi. Grazie a un tavolo tecnico permanente interistituzionale, emanato un nuovo decreto interministeriale, il n. 853 del 12 novembre 2020, con il quale si renderà possibile provvedere all'assegnazione delle risorse FIS anche per il prossimo triennio. Questo provvedimento, anche se non completa il panorama degli interventi che il Ministero intende adottare in tema di diritto allo studio, ha contribuito a superare le criticità esistenti, consentendo - da un lato - di evitare ritardi (oggi l'erogazione dei fondi arriva con l'inizio dell'anno accademico) e - dall'altro lato - di poter dare il beneficio delle borse di studio alla maggioranza degli studenti che ne hanno diritto. Concludo rassicurando i senatori che, nonostante gli interventi citati abbiano consentito negli ultimi anni uno sviluppo del sistema del diritto allo studio in questi termini, è mia intenzione accelerare il processo di adozione di tutti i provvedimenti richiesti dalla normativa e e ricostituire il tavolo tecnico in materia di LEP, che è composto anche da rappresentanti del CNSU, della CRUI, della Regioni e degli enti locali, che può dare un contributo molto importante per una nuova bozza di decreto in materia di diritto allo studio.

Sappiamo che, per chi non ha nulla, poter studiare è tutto, soprattutto nel tempo, come quello che viviamo, in cui la rivoluzione tecnologica lega sempre di più il lavoro alla competenza. Poter studiare significa diritto alla competenza e quindi diritto al lavoro. Questa urgenza, in questi mesi, ci viene consegnata anche da dati. Ad esempio, noi sappiamo che in questo anno accademico la media degli esami svolti è tornata ai livelli pre-Covid; tuttavia questo è un dato fuorviante se letto male. Sappiamo infatti che la didattica a distanza ha accelerato le carriere di chi è in condizioni economiche, abitative e familiari favorevoli e forti, mentre ha rallentato o anche fermato tutti gli altri, tra cui anche coloro che beneficiano di una borsa di studio, il cui importo è troppo esiguo e non può far fronte all'enormità dello *tsunami* che ci ha colpito. Così come, signora Ministro, noi sappiamo - e concludo, Presidente - che la riforma del calcolo ISEE, in assenza di un adeguamento al rialzo, da parte del Ministero, dei valori per l'accesso alla borsa di studio può creare un cortocircuito nella battaglia che insieme stiamo facendo per contrastare quel vero e proprio diritto negato che è quello dell'idoneo non beneficiario. Chiunque abbia merito deve essere sostenuto nella sua progressione e nella sua possibilità di futuro: questo è decisivo

ma anche e soprattutto le carenze: la carenza più grave che abbiamo affrontato e che ancora affrontiamo è quella di personale sanitario e, quindi, anche di personale medico, di medici specialisti e di medici di medicina generale. Questa carenza è certamente legata ai tagli trasversali che ha subito il nostro Servizio sanitario nazionale, ma anche a un'errata programmazione. Lei prima ne parlava, Ministra: oggi abbiamo uno strumento importante per la programmazione, che è quella tecnostruttura che abbiamo istituito con un emendamento alla legge di bilancio 2019, che permette ad Agenas e all'Osservatorio delle scuole di specializzazione di programmare il fabbisogno di specialisti in base al fabbisogno di salute della popolazione. Speriamo che sia presto operativa. Questa pandemia ci ha anche mostrato come sia fondamentale e indispensabile rafforzare il territorio, mettendo in rete e facendo lavorare in *team* multidisciplinari i medici specialisti e i medici di medicina generale, perché dal territorio deve partire la presa in carico precoce dei cittadini. Oggi abbiamo uno strumento importante per porre rimedio a dette carenze: questo strumento è il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che stanzia ingenti risorse proprio alla riforma della medicina del territorio, partendo dalle case e dagli ospedali di comunità. Ma quali sono gli specialisti che andranno a lavorare in quelle strutture? In diverse università italiane esiste una scuola di specializzazione, che è la scuola di specializzazione in medicina di comunità e cure primarie, che - secondo un decreto del Ministero medici specialisti per operare proprio nell'ambito della medicina generale, dell'assistenza primaria. Eppure, oggi questi medici non possono operare come medici di medicina generale. Quindi, Ministra, le chiediamo tre cose: innanzitutto se il Ministero intende sollecitare il Governo affinché questi medici specialisti possano operare come medici di medicina generale; in secondo luogo, se il suo Ministero intenda aumentare i contratti di formazione specialistica e medicina di comunità e cure primarie; in terzo luogo, come valorizzare questi specialisti affinché possano essere d'aiuto per il raggiungimento degli obiettivi di salute del PNRR e rendere finalmente operativo il Piano nazionale della cronicità.

devo rilevare che la competenza primaria - come già sapete - in materia di definizione dei contingenti per tipologia di scuola di specializzazione, compresa quella di comunità e cure primarie, compete al Ministero della salute, legislativo n. 368 del 1999. Questa considerazione vale anche per i contenuti della formazione specifica dei medici di medicina generale, ma questo lo sapete già. Ciò premesso, intendo riconoscere che alla questione posta dai senatori occorra dare rilievo per alcuni profili di interesse anche del Ministero dell'università. Come ho avuto modo di dire, il Governo è impegnato in un maggiore accrescimento del numero di borse di studio di formazione specialistica, perché ciò corrisponde a una necessità e a una necessaria risposta strategica rivolta a rafforzare l'intero Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il territorio. In questo processo di accrescimento ritengo opportuno che vi sia un incremento del numero dei contratti riservati alle scuole di specializzazione, inclusa la medicina di comunità e cure primarie. E questo lo segnalerò al Ministro della salute. Quanto alla richiesta specifica sull'assunzione di iniziative tese a monitorare le modalità con cui i medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie vengono valorizzati una volta che accedono al Servizio sanitario nazionale e in che misura concorrono alla realizzazione del PNRR, voglio dare una rassicurazione che questi obiettivi saranno perseguiti sempre d'intesa con il Ministero della salute e nell'ambito prevalentemente dell'Osservatorio di cui ho parlato prima. Concludo sottolineando un punto che credo molto importante per il nostro Ministero, e cioè che in questa fase di trasformazione del Paese, dove si stanno dimostrando indispensabili gli investimenti sul capitale umano, dobbiamo fare di tutto per focalizzare gli interventi volti ad elevare il livello della formazione dei nostri giovani, in particolare se a ciò corrisponde anche un più generale benefico effetto sulle capacità del SSN attraverso la valorizzazione della formazione di professionisti che saranno chiamati a operare anche nella medicina territoriale.

i contratti di formazione specialistica, che - voglio ricordare - nel 2018, quando siamo arrivati in Parlamento, erano appena 6.200, mentre oggi sono 13.400, e quindi sono più che raddoppiati. A questi si aggiungono i 3.000 di formazione in medicina generale. Quindi, la quasi totalità oggi dei medici che si laurea riesce ad avere ad avere un contratto di formazione specialistica. Oggi le abbiamo chiesto di questa specialità perché si tratta degli unici specialisti che non possono operare in tutti gli ambiti in cui vengono formati. Si formano in medicina generale. E questo e tecnologica (MURST) del 1996; lo ribadisce il decreto interministeriale del 2015 e anche la Direttiva europea del 2005 riconosce i requisiti per operare nella medicina generale e nella medicina territoriale a questi specialisti e, quindi, si tratta di un vero e proprio *vulnus* normativo che - a nostro avviso - va colmato.